gli interventi dei senatori Manzione e Mele che chiedevano una diversa organizzazione dei nostri lavori con riferimento ad alcune iniziative politiche, il Presidente del Senato ebbe a dire che nessuno modifica dei lavori del Senato può essere prevista se non con riferimento a congressi di partito. Io condivido questa impostazione che fa prevalere il dato istituzionale sul dato politico. Sento dire che anche domani mattina sono previste votazioni in Aula e come sempre faremo il nostro dovere. L'occasione mi è grata per sottolineare che credo questa sia una risposta alla mia protesta, avanzata nella seduta del 6 febbraio, quando il Presidente del Senato dichiarò che la discussione dei disegni di legge sul disagio abitativo sarebbe stata rinviata al giorno successivo per un impegno politico. Poiché anche in quel caso si trattava di una riunione di corrente di un partito, mi fa piacere che sia ripristinato il principio istituzionale; che la decisione di oggi sia scolpita in caratteri solidi perché non ci devono essere figli e figliastri.

La fabbrica della De Longhi - la nota industria di elettrodomestici - come lei forse saprà, è andata completamente in fumo.

a parte tutti gli interventi di protezione civile che sono in atto per salvaguardare la salute dei cittadini di Treviso e delle zone limitrofe, c'è un altro fatto estremamente grave: da domani mille dipendenti non avranno più un lavoro perché la fabbrica è completamente bruciata; non ci sono più neanche i muri, come si potrà vedere anche dai servizi giornalistici. Vorrei quindi che si facesse parte diligente nei confronti del Governo perché abbiamo sentito più volte parlare di vari tesoretti a disposizione dell'Esecutivo per le esigenze più varie. Ebbene, io penso che, al cospetto di una sciagura di questa portata portata (apro una parentesi perché mi hanno appena comunicato che su Treviso si sta sviluppando una densa nube di diossina il che è particolarmente preoccupante, non vorremmo si verificasse una nuova Seveso),

Signor Presidente, vorrei sottolineare che la mia non è assolutamente una questua, ma soltanto una necessità per il mio territorio e per tutta l'Italia.

si è trattato di uno *scoop*; per quanto concerne noi senatori e deputati, si è trattato di prendere contezza di una direttiva che il Presidente del Consiglio avrebbe dato ai propri Ministri, una direttiva gravissima

perché nella direttiva vi sarebbe scritto che i Ministri sono invitati a procedere per via amministrativa e a non presentare a causa delle difficoltà nell'approvazione. È il primo caso, almeno per quanto mi riguarda, in tanti anni che sono in Parlamento, che un Presidente del Consiglio dà una direttiva di questo tipo. Oltretutto,

che il Governo e il Presidente del Consiglio, nell'arco della giornata, l'avrebbero smentita, tanto mi pareva grave. Ma alle ore 17,10 del pomeriggio

ciò che dovremo fare, perché non riteniamo assolutamente possibile che questo possa accadere in un Paese democratico come l'Italia.

Va da sé - di questo informerò il presidente Marini - che ogni iniziativa che tendesse a limitare - semplicemente a limitare - le facoltà e le prerogative del Parlamento (in questo caso del Senato) verrà prontamente e con grande fermezza respinta dalla Presidenza del Senato.

negli stabilimenti del gruppo De Longhi, incendio che ha colpito, oltre ad un magazzino, due unità di produzione. Le preoccupazioni si rivolgono alla nube tossica che in questo momento si muove sopra la città (lo stabilimento è infatti ubicato nell'area urbana) e alla garanzia del reddito per i lavoratori, una parte dei quali, almeno, da domani non potrà continuare la propria attività lavorativa a causa della distruzione di queste parti dello stabilimento del gruppo.

Signor Presidente, mi associo a quanto già dichiarato dagli onorevoli colleghi eletti nella Provincia di Treviso, come la sottoscritta. Mi è stato riferito che a questo momento non ci sono feriti, ma che preoccupa la nube che si sta diffondendo; è già stato allertato il nucleo batteriologico e chimico della Protezione civile. Quindi, anch'io, esprimendo la massima preoccupazione per la salute dei cittadini della città e della Provincia di Treviso, chiedo che siano assunte le più dettagliate informazioni, che il Senato sia tenuto aggiornato e che siano prese tutte le iniziative utili salvaguardare la salute della popolazione. Esprimo, altresì, il massimo della solidarietà dell'azienda, ma anche a tutti coloro che, anche a rischio della propria incolumità, stanno lavorando per cercare di fare il possibile a favore della popolazione.

proposta di modifica dell'emendamento del Governo che introduce una copertura diversa da quella presente nell'attuale testo.

In via del tutto informale, io posso dire che, se il Governo depositasse formalmente la proposta di modifica del suo emendamento, il parere della il parere della 5a Commissione su tale emendamento rimarrebbe certo contrario senza riferimento all'articolo 81, ma si tratterebbe di una contrarietà decisamente meno rilevante di quella che avevamo formulato sul testo originario. Permarrebbero cioè dei problemi, ma non così seri e gravi come quelli che avevamo intravisto e valutato ci fossero a proposito del testo originario. Non so come si debba procedere formalmente; io questo sono in grado di dire, sulla base di quello che, per adesso, ho potuto prendere in esame. Forse qualche minuto di sospensione potrebbe essere la soluzione più ragionevole, ma può darsi che questa non sia del tutto idonea. Veda lei,

Presidente, mi scusi, io non conosco nel Regolamento pareri informali. Se il Governo ha un'altra copertura da presentare, non c'è altra via che la Commissione bilancio si riunisca e ne discuta; non riesco a capire come la Commissione possa formulare un parere preventivo. Se il Governo presenta un'altra copertura, la Commissione bilancio dovrà riunirsi ed esaminare la nuova copertura. Non vedo altra via. Signor Presidente, la situazione è abbastanza anomala. Noi abbiamo un emendamento da votare; normalmente, quando c'è un emendamento, lo si vota. Quell'emendamento - come abbiamo detto - presenta gravissimi problemi di copertura.

(che oggi, con un ravvedimento parziale e tardivo del Governo stesso, si tende a ridurre), l'opposizione mostra un senso di responsabilità particolare

riformulato nella copertura che il Governo ci ha detto intende presentare. Ci pare importante sottolineare tale questione, signor Presidente, perché il nostro atteggiamento assolutamente responsabile nei confronti di un rimedio che noi riteniamo tardivo e parziale, che noi proporremmo in forma ancora più radicale, ma che comunque si presenta come un *vulnus* gravissimo alle norme di contabilità pubblica, ci induce ad accedere alla richiesta fatta dal presidente Morando e quindi a derogare un po' al Regolamento del Senato, che prevede, viceversa, la

Signor Presidente, il Governo riteneva, nel momento in cui ha presentato un'ipotesi di copertura, che la stessa potesse essere considerata pienamente rispettosa delle norme. Allo stesso tempo, però, prende atto e rispetta l'autorevole parere dato in seguito all'esame approfondito - come di consuetudine - della 5ª Commissione, durante il quale il Presidente della Commissione stessa e autorevoli rappresentanti sia della maggioranza che dell'opposizione hanno sollevato, per usare un eufemismo, delle perplessità circa l'adeguatezza della forma tecnica di copertura dell'emendamento stesso. Quindi, nel pieno rispetto del parere formulato dalla 5ª Commissione, il Governo ritira l'emendamento in

chiesto eventualmente al Governo di precisare. Abbiamo svolto una riunione informale: bene ha fatto il senatore Boccia a chiedere una formalizzazione,

la nostra parte politica ritiene fondamentale che si mantenga un provvedimento, sul cui merito anche l'opposizione è d'accordo, che contribuisca ad eliminare i *ticket*. Pertanto, signor Presidente, le ribadisco la richiesta di sospensione perché riteniamo fondamentale votare un provvedimento che elimini i *ticket* almeno nella misura proposta dal ministro Turco. Invitiamo, quindi, il Governo a non ritirare l'emendamento e a permettere, con mezz'ora di sospensione, un approfondimento. Pur condividendo in astratto il percorso prima previsto (riunione della Commissione bilancio), oggi, di fronte ad un fatto politico nuovo, che è il ritiro dell'emendamento da parte del Sottosegretario, vi chiediamo una sospensione con un fine esplicito: poter salvare questa parte del provvedimento, la tendenziale abolizione dei *ticket*, che ci sembrava qualificante affinché non soltanto si tamponassero i *deficit* di alcune Regioni con un concetto di solidarietà del sistema sanitario, ma si desse anche un segnale.

come rappresentante dell'opposizione, ma anche come membro della 5a Commissione, fatico a comprendere di che cosa stiamo discutendo. Se ho capito bene, non si può procedere ad una sospensione per riunire la Commissione perché non c'è più l'emendamento a cui dobbiamo appostare una nuova copertura,

Presidente, non voglio, per carità, insegnarle alcunché, credo però che, stante l'importanza dell'emendamento 1.0.200 e stante il nostro Regolamento, dovrebbe prima verificare se qualche senatore in Aula desidera farlo proprio.

avendo seguito fin dall'inizio con attenzione questa vicenda, ritengo difficile che un emendamento del Governo, che era corredato da relazioni tecniche plurime (naturalmente, secondo noi, tutte non soddisfacenti, come si è dimostrato) e che era stato oggetto di un ragionamento assai complesso all'interno della Commissione bilancio, possa essere fatto proprio da un senatore. Credo che

tuttavia, sussiste un altro problema: la circostanza che il Governo ritiri un emendamento, a fronte di una richiesta di sospensione per verificare la possibilità di appostare una diversa copertura, non impedisce né a me, né ai colleghi di Rifondazione di far proprio l'emendamento; rende, però,

La Commissione bilancio pudicamente ha espresso un parere contrario senza riferimento all'articolo 81, ma sta di fatto che l'emendamento copriva una spesa corrente con soldi in conto capitale.

ad introdurre un emendamento che porterebbe a caducare il decreto. Se il Governo non è riuscito a trovare una copertura decente, non credo si possa trovare così, in qualche minuto. Caldamente raccomanderei all'Aula, visto che non c'è riuscito il Governo, che mediterà eventualmente una migliore copertura alla Camera, di ritenere ritenere chiusa la vicenda. Il Governo ha ritirato l'emendamento. Nessuno lo ripresenta in via pratica perché sarebbe un suicidio verso questo provvedimento e concludiamo il suo esame. Credo sia la strada migliore,

Lascio perdere gli effetti paradossali di questa situazione. Non è la prima volta che vediamo un Governo confuso. Abbiamo visto confabulare; abbiamo visto il ministro Turco probabilmente

anche il *deficit* di quelle Regioni. Quindi, credo che si debba fare ogni sforzo per eliminare questa palese iniquità da un decreto che è già palesemente iniquo. Quindi, da parte nostra siamo favorevoli affinché si riesca a trovare un'eventuale copertura.

è evidente che ci troviamo in un momento dove dire che c'è qualche equivoco è il meno che si possa fare. La richiesta di sospensione dei lavori formulata dal collega Sodano, secondo le procedure, è giusto che sia considerata dall'Assemblea e, per quanto ci riguarda, siamo favorevoli, soprattutto se serve a fare chiarezza sul valore dell'emendamento, sulla sua quantificazione e sulle eventuali coperture. Tuttavia, signor Presidente, è da evitare una sospensione se questa non serve.

inoltre; abbiamo avuto un parere contrario anche su un subemendamento. Signor Presidente, il Governo ha formulato la sua posizione adeguandosi a quella della Commissione,

per sospendere i lavori dell'Assemblea: si passa al voto sull'emendamento che un Gruppo ha fatto suo. Non ritengo che si debba riaprire una discussione in Commissione su un fatto che è usuale in qualsiasi Parlamento, non soltanto italiano ma del mondo, a meno che

Non vedo per quale motivo si debbano sospendere i lavori: si passi al voto e vediamo se il Parlamento, anzi, l'Aula del Senato redime questa controversia tra un Gruppo della maggioranza ed il Governo.

tecnica di copertura (e questo è stato anche l'esordio del mio intervento immediatamente precedente). Allo stesso tempo, il Governo vuole rispettare gli autorevoli pareri espressi dai membri della 5ª Commissione, a iniziare dal

in merito alla forma di copertura dello stesso emendamento: esclusivamente per rispetto del parere formulato dalla 5ª Commissione, dunque, il Governo ha ritirato l'emendamento 1.0.200. Dopodiché, atteso che l'emendamento stesso è stato fatto proprio da un altro senatore,

L'emendamento che viene riproposto è esattamente conforme alla proposta inizialmente formulata dal Governo; quindi, anche per un banale principio di non contraddizione, è evidente che il parere non può che essere favorevole. *(Applausi dal Signor Presidente, non capisco se il Governo ha rispetto per il Parlamento o ha fatto polemica con esso, perché altrimenti le questioni si pongono in maniera nettamente più grave.

Se il Governo ha rispetto, allora, coerentemente, ha ritirato un emendamento che sa bene avere un *vulnus* non profondo, ma lacerante, con la contabilità pubblica:

Commissione l'ha rinviato per trovare un'altra copertura e ne ha fatto circolare un altro informale, con una copertura ulteriore.

ad accettare, perché allora andava messo in votazione; e l'opposizione ha accettato la proposta di sospensione. A fronte di questo, il Governo dichiara di voler ritirare l'emendamento, dando così una visione politica condivisibile o meno (da noi non condivisa sul piano del merito, ma su quello della copertura, perché egli ha ammesso il *vulnus* lacerante della copertura sulla quale, se vi si dovesse dar corso, intenderemmo non continuare, ma cominciare il discorso). Infatti, a lei, signor Presidente del Senato, spetterà il compito di riferire al Presidente della Repubblica, che sul decreto-legge

le cose, chiedendo a lei, signor Presidente, garbatamente, che di questo sia fatto cenno esplicito nel messaggio al Presidente della Repubblica. Infatti, ove voi vogliate continuare a discutere di questo emendamento, porteremo gli esempi

le parole del Sottosegretario, oltretutto, abbiano anche spiegato correttamente l'atteggiamento del Governo.

a considerare l'opportunità di avere qualche minuto che ci consenta di verificare quale sia la strada migliore per uscire dalla situazione nella quale ci siamo infilati.

l'introduzione di quei *ticket* disposti dalla finanziaria viene eliminata per la seconda parte dell'anno. I pronunciamenti che vi sono stati in questa sede sul punto ci possono consentire di dire che l'Assemblea del Senato è unanime attorno alla positività di questa disposizione. Abbiamo sollevato in Commissione bilancio un serio problema sulla copertura di questa norma. Dopodiché non certo, senatore Castelli, in sede formale - lo avevo del resto detto chiaramente - ma in una discussione informale che a volte, lei sa, serve a preparare le decisioni formali, avevamo anche esaminato un'ipotesi di copertura alternativa a quella contenuta nel testo del Governo che naturalmente presentava a sua volta problemi di coerenza con la legge di contabilità, a mio avviso decisamente inferiori rispetto a quelli che presenta la proposta originaria del Governo. Allora, signor Presidente, prendo atto di quanto è accaduto, della decisione del senatore Sodano di fare proprio l'emendamento ritirato dal Governo, di quanto il Governo adesso ha detto sul parere che darebbe sull'emendamento a questo punto non più d'iniziativa del Governo, ma del senatore Sodano. Le chiedo formalmente, a mia volta, anche se il senatore Sodano ritira la proposta, di avere invece qualche minuto di tempo perché, per esempio, potrei decidere - e la prego di consentirmi di farlo anche se so che il Regolamento non è perfettamente tale da consentirmelo - di presentare assieme ad altri senatori un subemendamento all'emendamento Sodano, che ne cambia la copertura. Credo che, data la discussione che abbiamo sviluppato, sarebbe interesse generale consentire un'operazione che potrebbe rendere l'emendamento approvato meglio

di presentare un eventuale subemendamento solo per l'aspetto di copertura, tenendo conto di quello che dice il senatore Azzollini. Secondo me, in questo modo, potremo determinare

gli sforzi fatti in questo momento per risolvere la questione, ma il Regolamento parla chiaro. Il senatore Morando non me ne voglia, ma non ha alcun titolo per presentare emendamenti, a termini regolamentari. Gli emendamenti in questa fase possono essere presentati dal relatore, che non c'è, o dal Governo. Se il Governo vuole presentare un emendamento dietro suggerimento informale

Non capisco tutti questi strani contorcimenti. Se avessimo scelto questa via maestra, probabilmente adesso avremmo già votato, anziché essere rimasti incartati per un'ora a discutere.

Allora, comprendo quanto ha detto il presidente Morando, però vorremmo capire se questo è un percorso reale oppure se tra poco sarà di nuovo un percorso un percorso accidentato. Non siamo pregiudizionalmente contro la sospensione; vorremmo però capire cosa significa effettivamente e a quale obiettivo si vuole arrivare in caso di sospensione.

Signor Presidente, comincio dalla riformulazione della norma di copertura da parte del senatore Sodano, che, in sostanza, ha lasciato il primo comma esattamente com'era nella proposta originaria ed ha modificato il secondo comma, che reca la copertura dell'onere di 350 milioni di euro. In base all'articolo 100 del Regolamento e sulla base della discussione che già abbiamo svolto in Commissione bilancio a proposito della copertura precedentemente appostata dal Governo al suo emendamento,

troveranno nella riformulazione tagli agli appostamenti dei Ministeri. Bene, così come appare evidente, si tratta di tagli che sono assolutamente reali oggi, ma si tratta di somme che sarebbero state effettivamente spese in una fase successiva dell'anno; pertanto, avendo a base l'operazione dell'assestamento, sarà possibile naturalmente riappostare tutte queste risorse, in maniera tale che si possano ricostituire le disponibilità nei fondi che oggi sono qui coinvolti. Di conseguenza, lo dico ai colleghi, non dovrebbero esserci problemi creati da questa norma alla normale gestione dei fondi

vorrei sapere quale sia la fonte che ha consentito di modificare un emendamento a seduta già iniziata, dal momento che il Governo non lo ha fatto e il relatore non c'è. L'emendamento 1.0.200 (testo 2) è una riformulazione di un emendamento di cui è diventato titolare il collega Sodano: è quindi suo diritto riformularlo e potestà della Presidenza ritenerlo un nuovo emendamento o una riformulazione. Trattandosi di una modifica che interviene sulla copertura,

*(FI)*. Signor Presidente, mi soffermerò poco su questo subemendamento, analizzerò soprattutto gli aspetti di copertura, perché più interessante è la formulazione fatta dal senatore Sodano, sulla quale potrò intrattenermi più tardi. Questo subemendamento si limita a fare un'operazione che credo meriti l'approvazione di tutta l'Assemblea.

presenta molti aspetti negativi, pur essendo certamente migliore di quella precedente (su questo non ci sono dubbi, ma vorrò discuterla nel merito e nel metodo), non si comprende perché questo *ticket* non lo si

lo riduce ad una cifra assolutamente esigua rispetto a quella precedente, seppure onerosa per i cittadini: a questo punto è logico e coerente togliere, con altri 150 milioni di euro, l'intero *ticket*. Credo quindi che votare questo subemendamento sarebbe per l'Aula un un atto di tutta ragionevolezza. Per di più, quell'emendamento reca una copertura sfrondata da alcune sue voci che agli emendatori non paiono assolutamente opportune e per questo credo che a maggior ragione si possa votare. Ai colleghi di Rifondazione Comunista e ad altri che con

ferme restando alcune questioni di copertura che sono molto più rilevanti nell'emendamento presentato dal senatore Sodano e sulle quali mi riservo di discutere, credo che questo subemendamento possa essere tranquillamente accettato.

sono intervenuto per sottolineare francamente l'assurdità e la schizofrenia della posizione del Governo, che si dichiara favorevole a ridurre da 10 a 3,5 euro il *ticket*, ma contrario a ridurlo a zero. Faccio presente al Governo che i soli costi amministrativi del *ticket* sono valutati come ben più onerosi dello stesso *ticket* a 3-3,5 euro. Quindi, dal punto di vista finanziario, l'azzeramento del *ticket* costa meno che non limitarsi alla sua riduzione da 10 a 3,5 euro.

e legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Paesi in via di sviluppo): 320 milioni di euro. Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 50,

La seduta è ripresa.

viene individuata nella legge sui Paesi in via di sviluppo per 320 milioni di euro;

ci siano occasioni in cui è necessario assumersi la responsabilità facendo un discorso di grande verità,

perché il *ticket* di dieci euro sulla diagnostica è una misura che vogliamo correggere. stato infatti il Governo a presentare una riformulazione che prevede la riduzione da dieci euro a 3,5 euro, in accordo con le Regioni, compatibilmente con la situazione di passaggio in cui ci troviamo.

esclude le famiglie monoreddito con figli a carico, quindi la riforma complessiva e l'eliminazione complessiva dei dieci euro avverrà nella prossima legge finanziaria. Questo è il nostro impegno; esso consente di coniugare assunzioni di responsabilità verso i cittadini, equità e anche compatibilità di bilancio, permettendo inoltre di rispettare il patto con le Regioni. Perché - guardate - senza la cooperazione istituzionale non si governa una cosa difficile come la sanità.

(da 10 a 3,5 euro), è stato presentato dal Governo, senza che nessuno di voi ce lo sollecitasse. Questa è la prova della serietà, del rigore e della coerenza che con cui stiamo lavorando. Questa misura avviene dentro una politica della salute che ha visto, in una manovra finanziaria difficilissima,

ha visto stanziare 2 miliardi per ripianare il debito del 2006, un'eredità che voi ci avete lasciato. politica che difende la sanità pubblica, chiedo responsabilità, di fare i passi che si possono fare oggi, insieme, tenendo conto anche della collegialità del Governo. Non posso infatti essere indifferente al fatto che annullare annullare il *ticket* significa trovare una copertura che mette seriamente in difficoltà i miei colleghi di Governo su temi cruciali

del diritto alla salute, della difesa della sanità pubblica e del rispetto nei confronti dei cittadini dico: per favore, facciamo il passo che oggi possiamo fare - ossia passare da 10 a 3,5 euro -, con l'impegno a cambiare tutto il sistema di compartecipazione, in nome dell'equità, nella prossima legge finanziaria.

che il Governo in qualche misura è stato costretto ad accogliere perché non era quello che aveva presentato all'inizio, reca la previsione che si riduce il *ticket* grazie a 50 milioni di euro che si tolgono alla ricerca sulla salute,

e di non sottrarre risorse a questi fondi. Questa è la sostanza politica. Capisco perché il Ministro è così arrabbiata. Non mi riusciva di capire perché fosse così arrabbiata.

sembrava che fosse contraria all'emendamento stesso, per cui non ho capito più niente. Ora, grazie alla sua richiesta di chiarimento, la questione è chiara. Noi voteremo a favore dei subemendamenti per un motivo molto semplice: questo provvedimento è assolutamente iniquo. Come abbiamo ormai sviscerato ampiamente questo pomeriggio, il provvedimento in esame va a premiare chi spreca e castiga sempre doppiamente quelli che invece sono virtuosi. Pagano il *ticket*, pagano la sanità, e in più pagano le sanità non virtuose delle altre Regioni. *(Applausi Allora, siccome i padani sono stufi di pagare per tutti, quantomeno non paghi più nessuno. Questa è la logica per la quale siamo convinti che questi emendamenti, e soprattutto i subemendamenti, andavano sostenuti. Quantomeno faremo un favore ai contribuenti padani, che almeno, forse, non pagheranno più il *ticket* per sé e per gli altri. *(Applausi Presidente, mi prenoto in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.0.200 (testo

Presidente, prendo atto della riflessione del ministro Turco, alla quale va riconosciuta una responsabilità ed una capacità di affrontare con determinazione un problema significativo. Tuttavia, caro Ministro, ci consentirà di sottolineare che lei è stata costretta ad intervenire per una sorta di vicenda kafkiana, che si è determinata tra il Governo che lei rappresenta e la maggioranza che esprime il Governo che lei rappresenta. Si è aperta per questa strada, al di là dei rilievi di ordine procedurale o regolamentare, una sana dialettica parlamentare, che ha evidenziato due questioni. Voi avete posto un problema relativo ad una parziale diminuzione di quel*ticket* che voi stessi avevate inserito in finanziaria e rispetto al quale avevate bocciato gli emendamenti che questo Gruppo ha presentato in sede di finanziaria. Potrei dire che avete recuperato, dopo qualche mese, una parziale sensibilità rispetto al tema. Lei interviene, paradossalmente, per dire di fermarsi a questo punto, in quanto non si è in grado di fare un ulteriore passo. E lo fa, caro Ministro, dimostrando da una parte responsabilità, ma, dall'altra, avvalorando l'emendamento presentato dalla maggioranza, che interviene tagliando su fondi relativi alle politiche sociali. Cioè, mentre parliamo della famiglia dei giovani e della ricerca, voi ci proponete un emendamento per una parziale decurtazione del *ticket* e lo fate pagare alle famiglie, alla ricerca e alle politiche giovanili! Lei doveva andare fino in fondo! La verità è che la sua responsabilità si è fermata rispetto alla capacità di dire che la sua maggioranza è irresponsabile nel fornire la copertura finanziaria in questo modo. E noi siamo intervenuti, in una sana dialettica parlamentare, dimostrando che siamo un'opposizione governante, per rimodulare le coperture e per dire che il *ticket* è meglio abolirlo trovando coperture tali che, come ha dimostrato lo stesso subemendamento del senatore Mazzarello, vanno ad incidere sul fondo per i Paesi in via di sviluppo, preservando però i fondi per la ricerca e la salute, per la famiglia, per i non autosufficienti e per le politiche giovanili. Sta emergendo la vostra sostanziale ipocrisia perché, mentre discutete di riforma del *welfare*, mentre presentate, a ridosso del *family* *day*, un provvedimento di propaganda per destinare il tesoretto alla famiglia, incidete in questo modo sulla famiglia, sulle politiche giovanili e sulle ricerche. Basta con le ipocrisie! Abbiamo svelato la vostra sostanziale propaganda, anche rispetto al fondo per lo spettacolo. *(Applausi dal Gruppo* *FI*). abbiamo presentato un subemendamento che è, appunto, responsabile. Mi auguro che in una sana dialettica parlamentare sia possibile che il Parlamento si assuma la sua funzione di protagonista e dica con chiarezza

nella sua replica e ciò perché non è abituata a confrontarsi con il Parlamento. Oggi si è discusso e si è fatto, signor Ministro, quello che in genere dovrebbe essere un corretto lavoro di confronto parlamentare. Questa sua foga polemica, questa sua aggressività, suggerisco di riservarle al salotto di "Porta a porta" quando si confronta con qualche avversario

a presentare un emendamento del Governo che taglia il *ticket* e poi toglie i soldi ai Fondi per la famiglia e al Fondo per i non autosufficienti? Questo è puro canagliume sociale, puro canagliume sociale, significa sostanzialmente provocare il Parlamento. Voi siete dei provocatori e quindi non siete moralmente abilitati a venire in Aula e fare la polemica contro un'opposizione che dice: un tesoretto: esiste un tesorone!». Esistono 38 miliardi di euro di entrate aggiuntive non previste; 38 miliardi di euro che possono essere impegnati per una politica sociale, per un *welfare* sano.

Presidente, in verità, le avevo chiesto di parlare dopo l'intervento del ministro Turco, per dirle che avrei ritirato il mio emendamento, perché l'intervento del ministro è stato molto forte, molto positivo impegni molto significativi che il Governo si è assunto. Credo dunque che di ciò vada preso atto, anche con un gesto come quello che sto compiendo. Siamo passati, in questa giornata, da un momento in cui, per problemi di copertura finanziaria, c'era addirittura un ritorno indietro rispetto alla decisione positiva e importante del Governo di scendere fortemente con i *ticket* fino a 3 euro; fino a 3 euro; in questo momento, siamo di nuovo nella situazione in cui questo passaggio molto importante e molto positivo è riconfermato, cioè il valore del *ticket* si abbatte e soprattutto c'è un impegno del Ministro che ha detto chiaramente questo *ticket* sarà eliminato, soprattutto con la finanziaria del prossimo anno. Io insisterei, però, per dire che a questo punto bisogna trovare le coperture finanziarie giuste per verificare se è possibile farlo anche prima, perché è chiaro che nel momento in cui va ad una diminuzione molto importante e coraggiosa come quella che il Ministro ed il Governo e i miei colleghi che hanno sostenuto l'emendamento propongono qui, c'è un problema forse di convenienza complessiva

una visita specialistica, nella stragrande maggioranza delle Regioni del Sud, viene rimborsata 17 euro, poco più del costo di un'ora di una badante a Roma, quando si paga il *ticket*, quindi se lo si paga per intero; voi con la finanziaria avete aggiunto 10 euro. Quindi, lucrando 10 euro su ogni visita specialistica, perché 17 euro li date allo specialista e 10 li incamerate. Ciò vuol dire che voi state riducendo qualcosa di più del *ticket.* Se voi invece pensaste che 3,5 euro è il costo del *ticket* totale, sbagliereste e sarebbe un'idiozia, perché per recuperare il *ticket* e per vigilare il costo è di 5 euro a persona. Quindi, siate consci del fatto che con la finanziaria stavate lucrando sulle visite che che pagava la gente comune e che comunque con questo emendamento state solo riducendo a 3,5 euro una cifra iniqua, cioè stavate guadagnando sulla sofferenza della gente. Non usate più certi timbri di disgusto di fronte ad un atto che è di giustizia e che vi fa solo onore, perché avete sbagliato nel passato.

votiamo contro l'emendamento della maggioranza perché siamo contrari a questa sorta di macelleria sociale che questa sera viene proposta. Avremmo voluto più coraggio da parte del del Governo e da parte del Ministro: visto che è stata capace di reperire ben 3 miliardi di euro, avremmo voluto uno sforzo aggiuntivo o sostitutivo per eliminare il *ticket*, una tassa iniqua che colpisce indiscriminatamente i cittadini italiani. Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento che è stato presentato e sottoscritto anche da noi, oltre che dal collega Azzollini, ma non voteremo l'altro emendamento che configura una riduzione parziale ed ingiusta e che comunque non

definanziando altre norme. Signor Ministro, vorrei richiamare le sua gentile attenzione sul fatto che lei dovrà rifinanziare queste autorizzazioni che oggi vengono ridotte.

dovrà assumersi l'impegno di rifinanziare queste norme, non con l'assestamento, come è stato detto, ma con vere e proprie nuove leggi. Altrimenti, questo emendamento presenta problemi. Noi abbiamo acceduto alla metodologia in considerazione, signor Ministro, dell'importanza del provvedimento.

Noi l'abbiamo modificata. Si trattava di altri 130 milioni di euro su 460 e avremmo ridotto unanimemente il *ticket*. Avremmo avuto un gran successo nei confronti dei cittadini. Signor Ministro, lei non è stata capace di gestire un successo che sarebbe stato del Parlamento intero, maggioranza e opposizione.

quindi è del tutto naturale che l'opposizione metta in evidenza che la copertura che è stata adottata per realizzare questo intervento di riduzione drastica del *ticket* istituito

e mi rivolgo ai colleghi della maggioranza, al Governo e anche ai colleghi dell'opposizione, in buona sostanza questo intervento di copertura che cosa fa? Realizza un taglio su alcuni fondi di Tabella C.

Quindi, al di là della propaganda, ci troviamo in presenza di un intervento che riduce alcuni stanziamenti di Tabella C, i quali, colleghi di maggioranza, possono essere facilmente ricostituiti. potrebbero esserlo se, ripensando meglio tale misura nella lettura che di questo decreto vorrà fare la Camera, si potrà trovare una copertura diversa; tuttavia, anche se questo non avvenisse - e io non mi auguro che accada

e annullare i tagli che adesso si apportano a questi fondi. A quel punto, con apposito provvedimento legislativo (il primo che capita), utilizzando le risorse appostate in assestamento, si potrà realizzare la ricostituzione di questi fondi. Quindi - lo dico ai colleghi di maggioranza possiamo votare con assoluta tranquillità questo emendamento, perché facciamo una cosa buona riducendo drasticamente i *ticket* e saremo in grado facilmente queste disponibilità esattamente tra un mese e mezzo. Non capisco perché dovremmo avere esitazioni nell'approvare esattamente questo emendamento che ringrazio il collega Sodano di avere ripreso

cosa rimane rispetto alle risorse che qui vengono distratte. Infatti, in assenza del Ministro degli esteri e di Gino Strada vengono tolti 50 milioni di euro per i Paesi in via di sviluppo; in assenza della senatrice Rita Levi-Montalcini vengono tolti 50 milioni alle spese per la ricerca; in assenza del ministro Bindi vengono tolti 30 milioni al fondo per la famiglia; in assenza dei ministri Ferrero o Bindi, per le rispettive competenze, vengono tolti 30 milioni dal fondo per i non autosufficienti;

superiori agli anni precedenti. Ora vediamo un'inversione di tendenza e sappiamo quanto è faticoso far investire nella ricerca il privato, soprattutto di fronte a un segnale che vede lo Stato rinunciare a 50 milioni di euro

Onorevole Presidente, innanzi tutto vorrei confermare quanto aveva già dichiarato il presidente della 5ª Commissione permanente, senatore Morando,

pari a 350 milioni di euro, per l'anno 2007, saranno reintegrate dal Governo con apposito provvedimento legislativo da predisporre dopo l'adozione del provvedimento di assestamento del bilancio, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge finanziaria per il 2007. Quanto al parere, intendevo ribadire il giudizio positivo politico sul primo comma, che è rimasto invariato, e rimettermi complessivamente all'Aula.

Presidente, mi scusi, ma non può essere messo in votazione questo emendamento per parti separate, slegando la copertura dalla disposizione di spesa,

signor Presidente, mi deve chiedere il parere sulla prima parte, e chiaramente l'emendamento è scoperto per una cifra molto ingente (quella esattamente indicata, cioè 350 milioni di euro). La votazione deve avvenire unitariamente, altrimenti sfociamo in una situazione assolutamente ingovernabile. Senatore Morando, a me sembra di essere stato estremamente chiaro, come lo è stato anche il senatore Salvi nella richiesta al Governo di una valutazione complessivamente favorevole o contraria o di una remissione all'Assemblea.

che qualcuno ci riferisca qual è il parere - obbligatorio per Regolamento - del Governo su questo emendamento!

però, la signora Turco, che è Ministro, faccia meno comizi ed esprima più pareri, per favore.

è stato fatto proprio da esponenti della maggioranza ma, per tentare di giungere ad una sua approvazione, temo che in quest'Aula si stia realizzando un po' un gioco delle parti sulla pelle dei più deboli.

chiedendo ai colleghi della maggioranza di fermarsi, di prendere atto del fatto che il loro Governo ha ritirato quella proposta perché non vi è ancora una copertura seria,

noi siamo un'opposizione responsabile ma non potremo mai macchiarci le mani nel votare a favore di una copertura che toglie i fondi ai deboli e a chi ha bisogno di essere curato Con questo non voglio fare polemica nei confronti di nessuno perché il Governo aveva compiuto un atto di grande responsabilità, aveva ritirato la propria proposta e noi avevamo preso atto di tale scelta responsabile. Mi auguro

del fatto che il Governo in quest'Aula, ritirando l'emendamento, aveva riconosciuto che al momento una copertura finanziaria accettabile sotto il profilo politico e tecnico non c'era. *(Applausi

capita talvolta che un'opposizione irresponsabile voti demagogicamente a favore di un provvedimento sottraendosi alle responsabilità della copertura. Credo non sia mai capitato nella storia di questo Senato che sia il Governo a dichiararsi favorevole ad un emendamento sottraendosi alle responsabilità di una copertura ... *(Applausi E AN)* ... che il Governo stesso evidentemente sente come un incitamento ad una guerra fra poveri capace di creare fratture all'interno della società per la incapacità di affrontare seriamente il problema. che oggi noi votiamo qualcosa che crea un buco nel bilancio dello Stato, ovvero se non lo crea va a danno della ricerca, delle famiglie, della cooperazione internazionale,

dice quanto poco rispetto si abbia delle leggi e della logica ma anche della dignità del Senato. Fate dopo il provvedimento per abolire i *ticket*, quando avrete capito in che modo lo sapete e potete fare. Non prendete in giro il Senato! Non scatenate una guerra fra poveri; non create delle condizioni che ci fanno un po' - lo ammetto - vergognare del nostro Governo.

Storace è stato ministro - che consenta al sistema di sopportare una cifra che ciascuno di noi ritiene equa

subito manifestate, al punto che in Commissione bilancio si è sollevata un'obiezione sulla copertura che il Governo forniva a sostegno di questa ipotesi. La Commissione bilancio avrà lavorato

molto consistente del Senato, maggioranza e opposizione, che addirittura insiste: vi è stata un'ora di discussione nei corridoi, tra di noi, perché si vada oltre il tetto dei 3,5 euro.

tanto più lo sappiamo, perché non devo ricordare ai colleghi che siamo alla prima lettura del provvedimento, che scade il 19 maggio. Dunque, se ciascuno di noi è davvero fermo in quel convincimento - gli italiani hanno percepito che dai 10 euro si deve scendere ai 3,5 euro - davvero si può pensare che non si disponga di risorse tra la Camera ed il Senato per riuscire ad elaborare, nel tempo che ci separa dalla data ultima di conversione del decreto, una copertura più opportuna?

ai direttori generali dei Ministeri interessati sono già arrivate telefonate che dicono di stare tranquilli in ordine al ripristino, al restauro delle competenze.

sentirsi caricato della responsabilità di trovare una copertura tra Camera e Senato, di qui al 19 maggio, che sia in grado di sollevarci da questo problema transeunte e assolutamente ovviabile, come ci hanno spiegato sia il sottosegretario Sartor che il chiudere questa giornata in maniera da dire agli italiani: «Guardate che vi abbiamo abbassato il *ticket* da 10 a 3,5 euro e che da questo risultato indietro non si torna». Presidente, poco fa, l'Aula del Senato ha respinto un emendamento che azzerava il *ticket* senza fare «macelleria

e anche oggi lo ha dimostrato. Infatti, in un dibattito come questo, non è possibile che il Governo dica: «Mi rimetto all'Aula». Ciò vuol dire che questo Governo non è più nelle condizioni di gestire la governabilità del Paese. Fosse la prima volta, pazienza, ma ciò avviene anche su provvedimenti che non hanno nulla a che vedere con la spesa. Mi riferisco, ad esempio, al modo in cui il Governo aveva presentato un provvedimento sui Dico solo qualche giorno il Presidente del Consiglio ha detto: «Non è più un problema nostro; è un problema del Parlamento». Con un Governo come questo voi, colleghi della maggioranza, svolgete il ruolo di parlamentari, di Ministri, di Sottosegretari, perché Ministri e Sottosegretari non sono più in condizione di svolgerlo. Questo è ciò che oggi è venuto fuori in maniera evidente dal dibattito. Allora, ministro Turco, invece di parlare con le colleghe e i colleghi senatori, prenda il coraggio a quattro mani e dica che il Governo questa sera non vuole continuare, ritira il provvedimento e lo ripresenterà quando avrà la possibilità di trovare un'intesa. Altrimenti, possiamo fare in modo diverso:

era stata proposta prima dal Governo e poi fatta propria dal senatore Sodano ed é stata discussa - me ne daranno atto tutti i componenti della Commissione bilancio - approfonditamente come elemento coessenziale a un equilibrio del provvedimento per il ripiano selettivo dei debiti che ci apprestiamo a votare. Al di là di ogni strumentalizzazione, vi è una copertura iniziale prevista sul Fondo di rotazione della legge n. 183. A mio avviso, si tratta di una copertura anch'essa credibile, sulla quale la Commissione bilancio non aveva espresso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81; essa aveva rilevato incongruenze. In particolare, il presidente Azzollini

Al di là di qualche battutina, quanto alla questione della copertura dell'emendamento Sodano, vi è un impegno preciso del Governo e, aggiungo, del Parlamento. Il Governo presenterà, dopo l'assestamento, provvedimenti che il Parlamento potrà e vorrà sicuramente votare. Quanto poi al massacro**,** vorrei far rilevare all'opposizione che essa ha votato la copertura dell'emendamento principale del senatore Mazzarello, che prevedeva esattamente gli stessi tagli, tranne qualche aggravamento. Stiamo allora ai fatti. Oggi e non domani va votata la riduzione dei *ticket*; questo Parlamento sia sovrano oggi e quando voterà, dopo l'assestamento, il pieno ripristino delle tabelle. Per favore, presidente Azzollini, non giochiamo, affermando prima che tutti vogliamo

Questi definanziamenti sono effettivi e non ci potrà essere bilancio di assestamento che li copra. dovrà coprirli con risorse nuove e dovrà venire in Parlamento per le risorse nuove che dovrà appostare per

vengano rifinanziati, ove il Governo ritengo di farlo, con nuove risorse *ad hoc*. Questi - lo ribadisco - sono definanziamenti effettivi. Quando e se il Governo riterrà di dover

Io ho fatto una proposta che mi sembrava andare nell'interesse della maggioranza, ma se qualcuno non vuol comprendere, vuol dire che il voto finale verrà rinviato a domattina. Prego, senatrice Rubinato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, volto a sanare situazioni di disavanzo nel settore sanitario di alcune Regioni, rientra in un'impostazione dei rapporti tra Stato e Regioni non più adeguata al mutato quadro istituzionale. La riforma del Titolo V, finalizzata proprio ad un capovolgimento dei passati assetti istituzionali, richiederebbe piuttosto una maggiore responsabilizzazione delle Regioni, con conseguente assunzione di responsabilità per le politiche e per le scelte attuate in ambiti attribuiti alla competenza regionale. La strada da perseguire sarebbe quindi quella dell'attuazione di un federalismo fiscale proprio per dotare tutte le Regioni degli adeguati strumenti finanziari. Ma, ancora una volta, prevalgono logiche centralistiche, con un intervento dello Stato volto a sanare le situazioni finanziarie disastrose di alcune Regioni. Lo Stato diventa paradossalmente il tutore di quelle amministrazioni regionali che hanno prodotto un maggior *deficit* sanitario, sollevandole di fatto da ogni responsabilità e, anzi, premiandole con il trasferimento di ingenti risorse finanziarie per il ripiano del disavanzo. Ciò rappresenta una grave iniquità nei confronti di quelle Regioni virtuose che hanno saputo gestire in modo oculato la spesa sanitaria, anche attraverso l'introduzione di imposte non popolari, ma necessarie per far fronte ad essa. La pantomima odierna sui *ticket* sanitari è emblematica delle assurde contraddizioni in cui versano questa maggioranza e il suo Governo. E poi, Ministro, non è accettabile che chi ha ben amministrato venga punito e chi ha scialacquato venga addirittura premiato. Vorrei precisare che non si tratta di distinguere e contrapporre Nord e Sud, perché le Regioni virtuose e quelle con gravi *deficit* sono presenti in ogni parte del Paese, sia al Nord che al Sud. Noi siamo semplicemente contrari a qualsiasi forma di ingiustizia e di sperequazione nei confronti di tutte le Regioni, e non condividiamo che considerevoli risorse finanziarie vengano utilizzate per rimediare a comportamenti irresponsabili piuttosto che per attuare interventi di cui il Paese ha certamente più bisogno. Davvero non riusciamo a capire perché i cittadini delle altre Regioni, soprattutto quelle che hanno saputo contenere la spesa sanitaria, debbano pagare i debiti di quelle Regioni che si sono gravemente indebitate non riuscendo a tenerla sotto controllo. Non è certo con i provvedimenti tampone che si risolve il problema della crescita della spesa sanitaria, che grava sempre più pesantemente sui bilanci sia delle Regioni che dello Stato. Occorre una riforma organica, tesa a riorganizzare il settore sanitario, ad adottare una revisione e razionalizzazione dei criteri di spesa, e soprattutto occorre una maggiore responsabilizzazione delle Regioni, con l'attribuzione di adeguati strumenti finanziari. Ciò non è solo necessario, ma anche doveroso per dare attuazione ai principi e alle disposizioni stabilite dal nuovo Titolo V della Costituzione. Signor Presidente, onorevole Ministro, ci dispiace constatare che questo provvedimento va nella direzione esattamente opposta; si indirizza infatti in quella dell'iniquità, della deresponsabilizzazione e dell'incentivazione di politiche di spesa inefficienti, che producono forti disavanzi che lo Stato continua a sanare dopo che questo è successo. Ed è per questo, signor Presidente, che l'UDC esprime il suo convinto giudizio negativo su questo provvedimento.

delle migliaia di piccole e medie imprese che forniscono servizi alla sanità), ed anche con una grande attenzione alle carte. Diciamo, con grande franchezza, che non ci appassiona il tema, che pure è stato agitato in quest'Aula, di un provvedimento che non dovrebbe essere emanato perché, in qualche misura, discrimina le Regioni tra loro. Sappiamo bene che un provvedimento del genere fu già assunto nel 2001. nel 2001. Guardando le carte, crediamo si debba prendere atto che questo provvedimento interviene in uno scenario completamente diverso da quello descritto dal centro-sinistra e dallo stesso Governo fino a che non sono arrivate in Commissione le note tecniche che ha favorito grandi incomprensioni e reso perfettamente plausibile la rigidità di una parte del Senato rispetto a ciò che veniva proposto. Alludo anzitutto alle cifre, che finalmente abbiamo sotto gli occhi. Queste cifre raccontano di disavanzi ben diversi da quelli che sono stati proposti, anche e soprattutto sulla stampa. Cito fra tutti il caso del Lazio. Finisce, oggi, la pantomima dei 10 miliardi di debito del Lazio; i debiti del Lazio, certificati dalla Ragioneria generale dello Stato, sono di 4 miliardi e 200 milioni (e la metà sono stati fatti nel 2005). Finisce anche un'altra storia, che è durata ed ha aleggiato: quella dei debiti fantasma, che esistono solo sugli stati patrimoniali. Oggi l'*advisor* nominato dal Governo ci dice che questi debiti potrebbero addirittura non esistere. Rimangono tuttavia in piedi altre grandi questioni, che forse il Governo avrebbe dovuto raccontare all'Aula. E allora, forse, si sarebbe potuto andare anche oltre l'astensione. Le grandi questioni sono quelle che riguardano i ritardi nel concepire un meccanismo strutturale più equo di riparto dei fondi sulla sanità, ritardi talora incredibili. Ho informato la Commissione sul fatto che a Roma, nella nostra Capitale, mancano all'appello 160.000 abitanti dalla quota capitaria, misteriosamente scomparsi nel censimento del 2001 e miracolosamente riapparsi, ma non ancora registrati dall'ISTAT, appena il centro-destra ha perso le elezioni regionali. Sono 200 milioni di euro l'anno, solo quelli, di quota capitaria, che moltiplicati per cinque anni fanno un miliardo di euro che va calcolato in questo disavanzo. Bisogna tener presente il ritardo con cui si è provveduto a dare alle Regioni che avevano un'alta presenza di extracomunitari la possibilità di assisterli, di contarli nella quota capitaria.

problema da affrontare è quello di uscire da uno schema puramente comunicativo e propagandistico, che in materia contabile non paga, ed affrontare alcuni nodi importanti. Da questo punto di vista il Governo ha perso un'occasione ha perso un'occasione anche nella qualità del dibattito e nello spettacolo che si è offerto a quest'Aula sulla questione del *ticket* e anche quella di evitare alcuni cattivi gesti, come quello di tentare di non pagare gli interessi ai fornitori, o peggio ancora di fare una legge per proibire di fare i decreti ingiuntivi... PRESIDENTE. Senatore Augello, la prego il Gruppo di Alleanza Nazionale ribadisce in Aula quanto ha già sostenuto in Commissione, cioè la propria astensione su questo provvedimento.

E allora, come si può chiedere a quest'Aula e al Parlamento di intervenire ancora su un argomento su cui siamo già intervenuti finanziando dei provvedimenti

Inoltre fino al 1999 erano presenti anche gravi problemi di *budget* nell'ospedale, in quanto non c'era nessuna forma di aziendalizzazione e gli stessi bilanci non erano proventi di

costruttiva che l'opposizione ha rappresentato con un subemendamento. Infatti, in una giornata in cui si approva la legge di conversione di un decreto‑legge che stanzia 3 miliardi di euro a sostegno di alcune Regioni in difficoltà si è stralciata un'opportunità, che sarebbe costata 150 milioni di euro, a fronte di un'abolizione del *ticket*, che è una tassa, come tutti abbiamo convenuto, assolutamente ingiusta. Credo che l'arroganza con la quale il ministro Turco ha voluto non prendere in considerazione le nostre proposte sia stata un errore da parte della maggioranza. Per questi motivi, il Gruppo di Forza Italia dichiara la sua astensione.

Signor Presidente, questo decreto ha il limite di mantenere la questione della sanità su un terreno rigidamente economico-finanziario, consentendo anche le affermazioni semplificate sino alla brutalità che ho ascoltato qualche minuto fa. Per l'esperienza che ho del Sistema sanitario nazionale per avere avuto responsabilità di governo di una importante Regione meridionale, vorrei ricordare a tutti il tema della copertura dei disavanzi è un punto di osservazione troppo limitato del sistema, che non si fa carico della diversità dei punti di partenza e della mancanza di unitarietà del Servizio sanitario nazionale. I disavanzi sono spesso non frutto di una inefficienza, ma di costi del sistema che derivano da gravi *handicap*: la mobilità passiva, le infrastrutture, peso abnorme di una sanità privata che è nata per le carenze del sistema pubblico determinano spesso sui bilanci regionali gravami insuperabili. insuperabili. Il luogo di intervento più corretto è la sede del riparto del Fondo sanitario, ove i criteri di indirizzo dovrebbero contenere, accanto a meccanismi matematici formalmente equanimi, meccanismi d'intervento per combattere gli elementi strutturali di debolezza. E bene ha fatto il Governo ad utilizzare la prospettiva dei Fondi comunitari per un intervento di programmazione che possa in qualche modo incrementare le infrastrutture sanitarie. Se c'è un limite nel provvedimento è che non si sottrae ad una logica ragionieristica che è stata ben presente anche nella vicenda del *ticket*, senza riuscire a coinvolgere unitariamente il Parlamento in uno sforzo comune che tenga insieme il Paese sul servizio essenziale della sanità. Il voto del mio Gruppo, allora, è un voto contrario, ma è un voto contrario con molta sofferenza, perché questo è un tema nel quale lo sforzo comune ci deve assistere per garantire a tutti i cittadini italiani eguaglianza eguaglianza di assistenza, in quanto anche i meccanismi punitivi contenuti nella crescita dell'IRAP o dell'IRPEF sono doppiamente punitivi per quelle Regioni meridionali che scontano condizioni di sviluppo economico e di reddito delle persone fisiche fortemente negativi. Ma questo meccanismo non è di questo Governo: è un meccanismo precedente che in qualche modo grava sul terreno del reddito di quelle Regioni che hanno condizioni di debolezza. Ecco cosa mi aspetterei da questo Governo e dall'intero Parlamento: che sulla sanità, per il valore civile di questo tema, ci fosse uno sforzo per far avanzare il Paese e per garantire a tutti i cittadini condizioni equanimi di assistenza.